Signor Ministro, abbiamo valutato di interrogarla sui fondi corposi che il Ministero ha potuto

come strumento di rimotivazione territoriale, di superamento anche delle differenze sociali delle persone e come strumento per fornire quei mezzi che, appunto, se culturali, sono anche democratici e positivi per l'occupazione. Sono 22,2 i milioni di euro che andranno alle 14 Città metropolitane e a progetti di inclusione e, da quanto abbiamo appreso, 700.000 euro saranno destinati al Comune capoluogo di ogni Città metropolitana, a cui si aggiunge una quota proporzionale sulla base della popolazione residente in quel Comune. Riteniamo che siano risorse veramente importanti, che verranno utilizzate anche per sostenere le attività dello spettacolo dal vivo nelle aree periferiche e che riguarderanno sia i soggetti già finanziati nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) sia gli organismi professionali che operano da almeno tre anni.

22,2 milioni di euro di maggiori risorse disponibili sul FUS 2021 per sostegno di attività di spettacolo dal vivo, in tutte le varie forme, nelle aree periferiche. È stato adottato un criterio di distribuzione, individuando le aree metropolitane, che ovviamente hanno maggiore di aree periferiche e maggiori problemi al loro interno, destinando una cifra fissa ad ogni area metropolitana e una seconda parte, pari a 12,2 milioni di euro, in base alla popolazione. Ciò comporta che

capoluogo delle aree metropolitane. L'idea attorno alla quale ragionare - e credo che da questo punto di vista possa essere un segnale molto importante - non è semplicemente

Sono assolutamente d'accordo che sarebbe positivo rendere lo strumento permanente, e questa è la volontà mia e del Ministero. Ciò dipenderà ovviamente dalle risorse che il bilancio metterà a disposizione del FUS per il prossimo anno. Mi piacerebbe - anche se la decisione, su mia proposta, passerà poi al Consiglio superiore dello spettacolo

è all'attenzione dell'intera Commissione cultura ed è diventata un progetto trasversale, che non appartiene più quindi solo ad una parte. Pensiamo che forse con questa proposta di legge potremmo aiutare proprio il percorso di stabilizzazione. Siamo effettivamente convinti che, a partire dalle aree periferiche delle città, individuando anche altri tipi di periferie nel nostro così complesso territorio nazionale, potremmo con la cultura davvero invertire un processo e produrre una efficace inclusione. Siamo

Signor Ministro, la decisione di pubblicare in rete le immagini dei vasi italioti della collezione Rizzon, in consegna al Museo nazionale di Matera in modalità accesso aperto, e quindi - leggo dal comunicato stampa del I febbraio gratuitamente per qualsiasi scopo, è stata presentata da certa stampa come un progresso, un atto di lungimiranza della direttrice, uno sviluppo senza precedenti in Italia per un museo nazionale, secondo il comunicato. Ed è così in effetti, perché la normativa di settore lo proibisce, come lei sa, Ministro. Quella scelta illegittima non solo viola il quadro regolatorio vigente, ma rischia anche di produrre un danno erariale pari all'entità dei canoni non riscossi. La direttiva UE 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi al mercato unico digitale è stata recepita in Italia con il decreto legislativo n. 177 del 2021, che inserisce l'articolo 32-*quater* nella legge del 1941 sul diritto d'autore, mantenendo per i beni culturali le disposizioni in materia di riproduzione di cui agli articoli 106 e 108 del codice dei beni culturali e del paesaggio. Per l'articolo 108, comma 1, del codice, è l'autorità che ha in consegna i beni demaniali a determinare - caso per caso - i canoni di concessione e i corrispettivi, avendo riguardo soprattutto per l'uso e la destinazione delle riproduzioni. Previa autorizzazione, sono invece libere le attività di riproduzione svolte a fini di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa nonché promozione della conoscenza del patrimonio culturale. Quanto alla direttiva UE 2019/1024, che regola il riutilizzo dei dati del settore pubblico, nel caso di istituzioni culturali pubbliche essa prevede espressamente la vendita di riproduzioni dietro compenso. Il legislatore italiano ha pertanto inserito nel decreto legislativo n. 36 del 2006 l'articolo 12, che include, tra i dati di elevato valore, quelli dei musei, delle biblioteche e degli archivi pubblici. Orbene, l'autonomia speciale di cui gode il Museo nazionale di Matera non consente alla direttrice di inciuciare con i suoi amici francesi, Ministro, e di violare la normativa italiana, né lo consente al comitato scientifico che dovrebbe supportarla. Non basta. Una fondata censura su correttezza e trasparenza della selezione non concorsuale che ha posto il funzionario architetto in questione, grazie a un comma 6, alla direzione del Museo nazionale di Matera, ha accompagnato l'ammissione alla registrazione della sua nomina da parte della Corte dei conti. Il Ministero l'ha bellamente ignorata pur di ribadire la scelta del direttore generale musei. Ora, quello tace e il segretario generale tace anche lui davanti alla liberalizzazione senza riguardo per le finalità delle immagini della collezione Rizzon. Ma l'indirizzo politico spetta lei, Ministro, e non all'avvocato Nastasi né al professor Casini o al professor Osanna, la nuova trimurti. Le chiedo come intenda esercitarlo per garantire il ripristino e il rispetto della legalità anche nel cosiddetto Ministero della cultura. PRESIDENTE.

Con riferimento all'interrogazione, riporto quanto la direzione generale competente del Museo nazionale mi ha comunicato. Il Museo nazionale di Matera ha concluso un accordo di valorizzazione con il Centre Jean Bérard finalizzato, nell'ambito di una valorizzazione dei beni culturali in custodia presso il museo, e in particolare delle collezioni ceramiche in età classica-ellenistica, alla realizzazione di campagne fotografiche. Tale accordo non prevedeva e non prevede oneri di alcun tipo per l'amministrazione, prefiggendosi l'unico obiettivo di diffondere la conoscenza dei menzionati beni attraverso attività di ricerca condivise, finanziate interamente dagli istituti. Il Centre Jean Bérard è responsabile di diversi programmi di ricerca con fondi pubblici nell'ambito della missione archeologica in Sud Italia, e si interessa in particolare di ceramiche, appunto, in epoca classica-ellenistica. La produzione di immagini digitali ha riguardato pertanto solo alcuni fra i pezzi delle collezioni museali di maggior rilievo e pertinenza nell'ambito del progetto di valorizzazione. L'articolo 108 del codice nel disciplinare i canoni di concessione dei corrispettivi di riproduzione di beni custoditi presso gli istituti museali, prevede che «Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate purché attuate senza scopo di lucro». L'attività di valorizzazione del patrimonio e di diffusione della conoscenza dell'arte magno-greca per mezzo di una campagna fotografica, portata avanti dalla direzione nazionale del Museo di Matera, rientra pienamente nell'ambito disciplinato dalla menzionata norma, in considerazione della finalità istituzionale degli enti coinvolti esclusivamente volta ad attività di studio e ricerca. Peraltro, sempre in ottemperanza dell'articolo 108, comma 4, gli istituti hanno stipulato una polizza assicurativa necessaria per scongiurare qualsiasi pregiudizio, anche meramente eventuale, ai beni cultuali di quel progetto, e la direzione ha sottolineato in ogni caso che la gratuità, prevista dall'articolo 108 per casi come quello in esame, non sia in alcun modo suscettibile di produrre un danno economico per l'amministrazione, ma che anzi possa avere ricadute positive in termini di valorizzazione dei beni che il museo detiene in consegna, anche sotto il profilo di promozione e divulgazione della loro conoscenza. Tuttavia, considerato il quadro normativo vigente in materia, sono in corso approfondimenti presso i competenti uffici ministeriali sui termini e sulle modalità del progetto Museo di Matera, all'esito dei quali saranno eventualmente adottate iniziative. PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Corrado, per due minuti. non posso dichiararmi soddisfatta nonostante la rassicurazione finale del suo intervento. Anzi, devo dire che rimango indignata come cittadina e rappresentante dei cittadini per la sua risposta. I direttori dei musei con autonomia speciale non sono proprietari dei beni demaniali che hanno in consegna e non possono disporne *contra legem*. Non può farlo neanche lei, né può permettere che altri lo facciano. Ciò che avete consentito all'architetto Mauro, già direttore tecnico a Pompei senza interpello, ossia di violare la normativa e farsene vanto, ma non mi sorprende più di tanto perché tutti loro, tutti i ragazzi venuti da Pompei, mentore il professor Osanna nei suoi diversi ruoli, fanno quotidianamente danno all'immagine del Ministero e alle casse dello Stato. La Corte dei conti contestò la chiamata di Gabriel Zuchtriegel nella irregolarissima segreteria di Pompei, perché era un allievo di Osanna e aveva pubblicato insieme a lui. Se aveste impedito quella chiamata, ci saremmo risparmiati sia lo scandalo del teatro di Elea-Velia, sia il museo Casa delle streghe in un budello ferroviario di fine Ottocento, finanziato per quasi otto milioni di euro, e abbiamo rischiato che l'eredità passasse direttamente alla Toniolo, poi dirottata in Sardegna. Oggi la stessa situazione l'abbiamo con Enrico Rinaldi, che da Pompei è passato alla Direzione generale musei e ora è stato nominato direttore del Parco archeologico di Sepino in Molise, appena istituito (anzi, istituito appositamente per farne il parco autonomo di Ales, dal direttore all'ultimo custode). Da quando avete reso nota la sua nomina, in rete non compare più alcun *curriculum* del Rinaldi e - soprattutto - non si trova più alcun atto che comprovi quanto asserito nel comunicato stampa del Ministero, cioè né la docenza universitaria, né gli incarichi di RUP e direzione lavori per conto del Ministero stesso. Ministro, si tratta non più di opacità, ma di distorsione sistematica della realtà per occupare posti chiave e crearne di nuovi con i ragazzi venuti da Pompei, cloni del superdirettore, sempre intento a celebrare la propria gloria e non solo nell'alto dei cieli. Cialtronerie...

perso il lavoro o siano stati costretti dagli eventi a reimpiegarsi in settori diversi dal loro. Sotto Natale le inevitabili restrizioni hanno impedito a quel settore di prendere qualche boccata d'ossigeno dovuto alle festività natalizie. In tutto ciò, il cosiddetto decreto ristori-*bis* è stato licenziato lo scorso luglio e il suo Ministero non ha ancora pubblicato il bando che consente agli impresari dello spettacolo di accedere a quelle magre somme. Le chiedo, pertanto, qual è la ragione di questo ritardo e se non sia opportuno anche rivedere le regole e la documentazione necessaria per poter accedere a questo contributo pubblico. Sono quanto di più lontano dall'idea di incentivare l'evasione fiscale, ma mi chiedo se abbia senso chiedere il rigido rispetto del DURC, e quindi della fedeltà fiscale delle micro aziende del settore dello spettacolo, che - giocoforza - in questi due anni

come il senatore Cangini sa, i danni che il settore ha avuto sono enormi e ad essi sono corrisposte molto risorse, che sono state utilizzate per tutti i settori dello spettacolo dal vivo, anche quelli che tradizionalmente non avevano mai avuto risorse pubbliche

a teatri e cinema di avere la normale funzionalità e, quindi, il normale accesso di pubblico, e ciò è avvenuto anche se si è registrato, in particolare nel settore del teatro e dei concerti, un ritorno molto più forte (più forte, purtroppo, del ritorno alle sale cinematografiche). Sono in fase di preparazione i bandi

desidero sottolineare che la previsione concernente il requisito della regolarità contributiva prevista dal DURC ai fini dell'accesso, da parte delle imprese che esercitano attività nell'ambito dello dello spettacolo, a ogni tipo di sovvenzione, contributo o premio statale, rinviene il proprio fondamento in una disposizione di legge primaria, e non in un atto amministrativo. I decreti ministeriali nonché i bandi sono tutte fonti sottordinate rispetto alla legge nel prevedere tale requisito e, quindi, non fanno altro che conformarsi come devono fare - alla norma primaria. Peraltro, facendo applicazione delle disposizioni normative in materia di DURC, il Ministero ha cercato di temperarle erogando i contributi anche in favore di quei soggetti che hanno provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva in epoca successiva alla presentazione della domanda e che, pertanto, risultavano in regola con il pagamento dei contributi previdenziali al momento dell'erogazione del contributo e non al momento dell'erogazione della domanda; ciò anche a seguito dell'invito dei predetti organi a trattenere dalle somme dovute dalle imprese sopra menzionate l'importo corrispondente al debito contributivo accertato. Alla luce di questo quadro, condivido il tema che in emergenza alcune misure dovrebbe essere allentate, ma ritengo, senatore Cangini, che serva un intervento legislativo e credo che sia il Parlamento l'unico organo che può evidentemente modificare quella norma, alla quale saremo felici di adeguarci, se modificata.

resta l'incongruenza del fatto che non sia stato ancora liquidato il secondo, che risale a sei mesi fa. Signor Ministro, tutti in quest'Aula e in quella della Camera ci stiamo ponendo il problema di come ristorare e rendere il dovuto onore a quei medici e infermieri che hanno curato e curano i nostri corpi in questa fase pandemica. Credo che dovremmo avere la stessa attenzione anche per quei musicisti, quegli attori e quegli impresari dello spettacolo che curano la nostra anima e alleggeriscono il nostro spirito, perché a mio avviso non rendono un servizio pubblico minore.

aperta nel corso del 2021, è stata la conseguenza di un periodo particolarmente lungo di condizioni meteorologiche, geopolitiche e di mercato eccezionali,

Il preoccupante aumento dei prezzi si è riverberato anche nell'aumento dei prezzi dell'elettricità in Italia ed è la causa principale del rincaro delle bollette di gas e luce, soprattutto determinato dal fatto che i prezzi del gas naturale sono aumentati addirittura del 660

41,8 per cento per quella del gas nel primo trimestre del 2022. L'impatto sulla spesa delle famiglie è evidentemente pesantissimo. La scelta degli Stati di perseguire obiettivi di lungo termine, come la decarbonizzazione dei sistemi produttivi e la mitigazione del surriscaldamento globale - da un alto - ha favorito gli investimenti nella generazione di energia da fonti rinnovabili, determinando quindi una netta espansione della domanda globale di gas naturale e gas naturale liquefatto, combustibili ponte nel processo di transizione energetica. Dall'altro lato, però, tale scelta ha disincentivato gli investimenti nella produzione di energia da altre fonti fossili, portando quindi alla necessità di interruzioni e riqualificazioni di infrastrutture chiave del gas. La produzione di energia elettrica in Europa inferiore rispetto al 2020, seguita da una diminuzione di centrali nucleari e dall'aumento dei prezzi del carbone, ha contribuito a intensificare le crisi energetiche; la mancanza di fornitura di gas verso l'Unione europea ha posto notevoli problematiche strutturali legate alla dipendenza interna per oltre il 50 per cento dell'approvvigionamento delle fonti del gas da un solo fornitore (la Russia), nonché i problemi che tutti conosciamo per l'attuale situazione fra quel Paese e l'Ucraina. Inoltre, il costo delle bollette per le aziende è pressoché raddoppiato e la situazione energetica in corso ha fatto emergere una serie di questioni e problemi strutturali, per cui occorrono interventi immediati, come lo stanziamento di risorse pubbliche per contenere il caro bollette. tutto questo, vorremmo sapere quali misure il signor Ministro ha posto in essere per aiutare le imprese che si sono trovate a fronteggiare perdite enormi a seguito del rincaro delle bollette e quali intenda adottare per il rilancio del sistema produttivo italiano; tutto ciò considerato, oltretutto, che giornalmente leggiamo sui giornali notizie di aziende costrette alla chiusura o al ridimensionamento della propria attività proprio a causa di questi

Il Governo è intervenuto in via d'urgenza ripetutamente, da ultimo con il terzo decreto-legge sostegni del 27 gennaio 2022, che, oltre ad agire nuovamente per cercare di ridurre e attutire l'impatto sulle bollette per le famiglie, si è dedicato anche giustamente all'impatto sul sistema produttivo, azzerando gli oneri di sistema a carico delle imprese in generale. Per quanto riguarda le cosiddette imprese energivore, ha parzialmente (e solo parzialmente) compensato i sovraccosti derivanti dal caro energia. Sono assolutamente consapevole che questa misura non è sufficiente. Credo che già domani, o comunque rapidamente, il Governo interverrà di nuovo cercando di prevedere o di replicare anche per il secondo trimestre le misure che abbiamo già adottato a gennaio.

i casi di autoproduzione dell'energia - per fare un esempio - che sostanzialmente risentono due volte l'incremento del prezzo del gas. È evidente che l'ammontare degli aumenti richiederebbe richiederebbe disponibilità finanziarie ben oltre quelle consentite dall'attuale strumento di bilancio. Molto faticosamente al Ministero dell'economia e delle finanze si sta cercando di costruire una dote finanziaria significativa; ma, a bilancio invariato, è evidentemente molto difficile dare una risposta compiuta e definitiva a questo tipo di fenomeno. Più complessivamente, guardando all'orizzonte di medio-lungo termine, è chiaro che dobbiamo fare determinati tipi di politiche. Quello che sicuramente possiamo fare oggi, in particolare sul gas naturale, è aumentare la produzione, gestire molto meglio lo stoccaggio e in modo strategico gli approvvigionamenti, anche se come è evidente - la dinamica a livello internazionale di tipo geopolitico ci crea qualche problema che non è esattamente nelle nostre disponibilità e delle nostre leve. Quello che Quello che dobbiamo fare è cercare di aumentare la produzione nazionale e in qualche modo introdurre dei meccanismi, che sono già allo studio e che credo e spero riusciranno a diventare norma a breve, di calmierazione di prezzo con riferimento a determinati settori produttivi. È un tipo di sfida che ci ci costringe ad agire in ottica di emergenza, ma che inevitabilmente induce l'Italia e l'Europa anche a una riflessione di medio-lungo termine che riguarda la sovranità strategica e anche l'autonomia politica dell'Europa e dell'Italia.

Sappiamo che le risorse attuali non bastano e che abbiamo bisogno di misure differenti. Confidiamo quindi molto nella sua attività e nell'attività del Ministero che lei dirige perché vengano attuate nell'immediatezza e non vengono rinviate. Di questi temi si parla veramente da tanto tempo, ma

*(FdI)*. Signor Ministro, questa interrogazione nasce sulla scorta di alcune sue dichiarazioni rilasciate alla stampa nei giorni scorsi, in cui lei ha testualmente affermato che il superbonus ha funzionato, ma sta drogando l'edilizia, mentre ci sono altri settori che vanno attenzionati, come l'*automotive*, dove il passaggio all'elettrico rischia di creare una ecatombe in termini occupazionali. Certamente lo scenario che lei delinea è serio ed è meritevole di attenzione, ma non capiamo francamente la finalità. Fino ad ora, da vent'anni a questa parte, il settore delle auto è stato sempre utilizzato come bancomat da parte dello Stato. Ora ci sembra di capire dalle sue parole che l'*automotive* ha bisogno di sostegni, ma non può riceverli perché è stato introdotto il superbonus. Noi non pensiamo che sia questo l'approccio da avere in detto caso. Il superbonus è stata una grande opportunità per il settore edilizio: prova ne è che ha favorito la nascita di migliaia di imprese, ha favorito la creazione di centinaia di migliaia di posti di lavoro ed ha generato importanti introiti per le casse dello Stato in termini di IVA, di Irpef, di Ires e di IRAP, che sono arrivati proprio da quei versamenti fiscali inerenti le migliaia di cantieri aperti nell'ultimo anno trascorso. Vede, signor Ministro, questo non lo diciamo noi di Fratelli d'Italia, ma lo dicono autorevoli studi di settore ed analisi fatte anche dai nostri uffici parlamentari del bilancio. Non vorremmo che dalle sue parole emergesse la volontà di favorire un settore che necessita giustamente di attenzione, ma a scapito di un altro che invece ha funzionato molto bene e che, al netto delle truffe che ci sono state, e che indubbiamente vanno contrastate con ogni mezzo, non merita lo stop che gli si sta imponendo in questi giorni, da quando è stato emanato il decreto-legge sostegni-*ter*, con l'ennesima modifica retroattiva che non fa che creare confusione, incertezza e frena gli investimenti da parte degli imprenditori onesti. Quindi, Ministro, con questa nostra interrogazione le chiediamo se può dare in qualche modo garanzie circa le iniziative che il Governo intende assumere per dare certezze a questo settore.

con migliaia di persone che perderanno il posto di lavoro. In quell'intervista io non ho contestato il superbonus come misura di politica industriale in favore del settore dell'edilizia, che ha funzionato

a chi potenzialmente guadagna 300.000 o 400.000 euro e ristruttura la terza o la quinta casa, secondo me, per il mio Ministero, c'è un problema. Io ho l'esigenza di richiamare il Parlamento e i colleghi del Governo che analoga attenzione e analoghe risorse devono essere destinate anche ad altri settori industriali, che oggi fronteggiano una crisi epocale.

Dopodiché spero che a brevissimo il Parlamento e il Governo dedichino altrettanta attenzione alle sfide epocali del settore dell'*automotive*, altrimenti saremo di fronte a una crisi epocale, nella produzione diretta e nell'indotto. Tornando al discorso del superbonus,

oggettivamente una situazione di blocco e di grave tensione nel settore, si rimedierà a brevissimo con un provvedimento di urgenza, che conterrà però anche altre misure per per normalizzare l'attività economica legata all'edilizia e al superbonus, ivi compresi - credo di poter anticipare - nuovi strumenti sanzionatori per reprimere ed evitare il sistema delle frodi. Dobbiamo contemperare quindi due opposte esigenze. La prima è l'esigenza di spingere il più possibile l'economia alla ripresa; a questo fine - l'ho detto nell'intervista e lo ribadisco adesso - ha avuto un ruolo fondamentale non soltanto il superbonus, ma tutto il sistema degli incentivi all'edilizia, perché direttamente si trasmettono all'economia nella fase della grande crisi. Ma oggi non possiamo pensare che il futuro industriale del Paese sia soltanto l'edilizia; è importante, ma c'è anche la manifattura, che ricordo, per quanto riguarda l'Italia, è la seconda manifattura d'Europa, dietro soltanto alla Germania. Non possiamo pensare a un'Italia che nel futuro non sia a presidio dei settori tecnologicamente più avanzati.

il superbonus per l'edilizia e bene l'edilizia, anche se dobbiamo in qualche modo limitare le cose sbagliate che ci sono, ma dobbiamo anche dedicare tanta attenzione a tutti gli altri settori industriali, che fino a questo momento non hanno ricevuto la medesima attenzione.

a persone che hanno 300.000 o 400.000 euro di reddito e a chi ha la quarta o la quinta casa. Intanto non funziona così, perché noi ci fermiamo all'abitazione principale e al massimo alla seconda abitazione. Ma io le posso anche dire che noi spendiamo

non ci convince. Abbiamo contezza del fatto che, per quanto riguarda la misura del superbonus, abbiamo dato risposte a migliaia di famiglie e a migliaia di imprese che rappresentano la spina dorsale del sistema economico del nostro Paese. Noi auspichiamo che

sindacato ispettivo riguarda la crisi aziendale della ACC Compressors, ex Zanussi Elettromeccanica, un'azienda storica situata nell'area di Belluno, fondata nel lontano 1960 e *leader* nella produzione di compressori per uso domestico. una questione a nome del Gruppo parlamentare della Lega, in particolare dei colleghi veneti Romeo, Candura, Fregolent, Ostellari, Pizzol, Vallardi, Zuliani - permettetemi - anche a nome del compianto collega Paolo Saviane che da quel territorio proveniva e che lo ha sempre rappresentato con grande spirito di servizio e passione. nel 2003 è stata ceduta da Electrolux a un fondo di *private equity* e nel 2009 è entrata in crisi finanziaria; nel 2013 è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria; nel 2014, il Ministero dello sviluppo economico ha aggiudicato la procedura di dismissione del complesso aziendale in favore del gruppo cinese Wanbao, dando vita alla società Wanbao-ACC;

hanno comportato un impatto significativo sui prezzi, tale da non poter ottenere un margine di contribuzione positivo; gli azionisti inizialmente hanno rispettato gli impegni assunti presso il Ministero dello sviluppo economico, ripianando le perdite di esercizio fino al 2019. Tuttavia, a marzo del 2020 la società ha chiesto la dichiarazione dello stato di insolvenza e, dopo l'accoglimento del ricorso nello stesso mese di marzo 2020, a maggio 2020 la società è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria; a maggio 2021 era stata avviata una procedura competitiva per la cessione del ramo aziendale, che aveva sollevato l'interesse dei principali operatori mondiali del settore, ma alla data di scadenza del 6 ottobre 2021 non è stata ricevuta alcuna offerta;

sono pervenute ufficialmente tre manifestazioni d'interesse. Si chiede in definitiva di sapere quali iniziative di propria competenza il Ministro interrogato intenda adottare al fine di individuare celermente il percorso più idoneo volto a garantire prospettive occupazionali e un rilancio produttivo dello stabilimento ACC di Belluno, in un'area caratterizzata da altre situazioni di crisi. il senatore Tosato per avere ripercorso storia e la vicenda di questa azienda: crisi, salvataggio con un'impresa cinese, che poi a sua volta è fuggita, portando via per cui l'azienda è ripiombata nella crisi, che è stata gestita secondo gli strumenti e secondo le procedure della nostra normativa. Grazie per aver richiamato il fatto che un'azienda non è semplicemente un valore economico; per un territorio essa è un dato anche culturale, proprio della cultura del lavoro di queste zone, con la passione che tutti i soggetti, enti locali, Regioni, sindacati, hanno manifestato nei confronti del Ministero per cercare di arrivare a una soluzione

abbiamo autorizzato l'aggiudicazione del complesso aziendale alla società SEST SpA, con sede a Limana, Belluno, la quale appartiene al gruppo italiano LU-VE, uno dei primi operatori mondiali nel settore degli scambiatori di calore d'aria e quotato nel segmento Euronext della Borsa di Milano. che nel 2020 ha registrato un fatturato consolidato di oltre 400 milioni di euro. La proposta vincolante di acquisto da parte della SEST SpA prevede in particolare la completa riconversione industriale del complesso aziendale al fine di ampliare la produzione di scambiatori di calore statici per banchi frigoriferi, condizionamento d'aria, pompe di calore, già presenti nel vicino stabilimento di Limana. Le procedure esperite sul mercato non hanno fatto emergere iniziative imprenditoriali per l'attività tradizionale, tipica della produzione e commercializzazione dei compressori per uso domestico. D'altro canto, come anche riportato nell'interrogazione stessa, la concezione del compressore per uso domestico impone produzioni in larghissima scala che non sono compatibili né replicabili nel nostro Paese. Questo primo ed importante passo è stato reso possibile grazie all'impegno di chi ha seguito la via della realtà e della concretezza, abbandonando percorsi che possiamo Questo caso è paradigmatico anche perché interviene - e di questo credo che possa andare orgoglioso anche quel territorio - un'azienda del territorio a salvare una situazione di crisi generata dallo scorretto comportamento di società multinazionali con investimenti di carattere predatorio, attuando però al

in tanti altri casi, dalla rivoluzione ambientale digitale, ci impone veramente di ragionare di fronte ai cambiamenti che si prospettano al sistema industriale in modo innovativo e flessibile. Tutti quanti, politica, parti sociali, associazioni imprenditoriali e sindacati, devono interpretare questa nuova fase, con le relative implicazioni strategiche, nel modo corretto per trovare soluzioni a beneficio dei territori e, in particolare, dei dipendenti e degli operai interessati.

La ringrazio e, a differenza di chi mi ha preceduto, non ho colto propaganda nelle sue parole, ma risposte concrete, utili al bene comune. Il settore manifatturiero e industriale è fondamentale per la crescita e il benessere di un Paese, come ha detto anche lei in un precedente intervento. Aziende collocate in territori montani e pedemontani vanno difese, rappresentando uno sbocco fondamentale per l'occupazione dei giovani di quei territori. L'alternativa è l'abbandono della propria terra in cerca di fortuna altrove, a partire dalle grandi città o verso l'estero per chi ne ha l'opportunità. Gli effetti della pandemia, il caro energie e la mancanza di materie prime stanno mettendo seriamente a rischio la tenuta del sistema produttivo dell'Italia, già in crisi in molti settori per ragioni di competitività. Il Governo e il Parlamento hanno il dovere di affrontare questa difficile congiuntura con grande impegno e unità di intenti. Siamo lieti che nel caso della storica azienda bellunese il Ministro stia riuscendo ad ottenere i risultati confortanti perché la salvezza di ogni singolo posto di lavoro significa salvare una famiglia da crisi profonde economiche, sociali e personali. Il compito che le è stato assegnato è gravoso, ma siamo sicuri che il Ministero dello sviluppo economico è in ottime mani. Il Gruppo Lega sarà sempre al suo fianco e a quello del Governo, in prima linea per difendere aziende e posti di lavoro. Crediamo ancora che all'Italia appartenga la cultura del lavoro convinti che l'Italia non possa abbandonare la propria vocazione di Paese industrializzato. Ognuno di noi deve fare la propria parte in questa direzione. In questa fase così difficile non potevamo stare a bordo campo a guardare e a criticare ciò che facevano o non facevano gli altri; sarebbe stata esclusivamente una posizione di comodo. Altri hanno fatto questa scelta; noi abbiamo scelto un percorso più difficile per noi, ma più utile al Paese. *(Applausi).*

*(M5S)*. Signor Ministro, i cambiamenti climatici e il degrado ambientale sono ormai una minaccia enorme per l'Europa e per il mondo. Per superare tali sfide, a luglio 2020 la Commissione europea ha presentato il *green deal* europeo, che trasformerà l'Unione in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, garantendo che nel 2050 non siano più generate emissioni nette di gas a effetto serra e che la crescita economica sia dissociata dall'uso delle risorse. Gli Stati membri pertanto sono impegnati ad affrontare i bisogni che il cambiamento epocale richiede rispetto ai nuovi stili di vita e ai modelli di consumo dei beni, che comportano necessariamente una trasformazione radicale dei processi con una forte spinta all'innovazione nei sistemi di produzione e di consumo. L'Italia, in risposta a tali sfide, tramite il Comitato nazionale per la transizione ecologica, si è dotata di un Piano per la transizione ecologica (PTE) che coordina le politiche in materia di raccordo con il *green new deal* europeo e il Piano PTE individua le azioni, le misure, le fonti di finanziamento e il cronoprogramma, nonché le amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure, articolate in otto ambiti di intervento previsti, per i quali verranno costituiti appositi gruppi di lavoro: decarbonizzazione, mobilità, qualità dell'aria, suolo, dissesto, risorse idriche, infrastrutture, biodiversità, il mare, la promozione dell'economica circolare, della bioeconomia e dell'agricoltura sostenibile. Un ruolo strategico, in coerenza con la pianificazione del PTE, è rivestito dal settore produttivo industriale che, per mantenere la propria competitività, dovrà adeguare i vecchi sistemi produttivi a nuovi modelli, fortemente innovativi e ambientalmente sostenibili. A tal fine, è necessario che lo Stato, attraverso misure e azioni di dettaglio, accompagni in questo passaggio storico il tessuto produttivo, in particolare i cosiddetti settori *hard to abate* e *automotive*. Attualmente sono disponibili alcuni strumenti per sostenere interventi strutturali rivolti alla decarbonizzazione e alla riconversione, con risorse disponibili dall'Emission trading scheme (ETS), dal PNRR, dal Piano di transizione 4.0 e dal Fondo per la decarbonizzazione previsto nell'ultima legge di bilancio. Tuttavia, occorre velocizzarne l'applicazione, introducendo e sostenendo con convinzione nuovi strumenti e innovazioni tecnologiche, in particolare dirette a sostenere l'autonomia energetica delle attività produttive, attraverso la creazione di configurazioni, come le comunità energetiche e l'autoconsumo diretto, che permettano di ridurre i costi dell'energia. Le chiedo di sapere come ritenga di sostenere il processo di innovazione in ottica di transizione ecologica e, in particolare, quali misure intenda adottare per accompagnare in tale percorso i differenti comparti industriali, assicurando competitività e sostenibilità ambientale delle imprese.

strategico di come il nostro Paese possa affrontare la grande sfida della rivoluzione ambientale e della rivoluzione digitale e la sua traduzione nel nuovo sistema industriale ed economico del Paese. l'attività cui si dedica evidentemente il Piano nazionale di ripresa e resilienza con interventi di natura trasversale in cui il Ministero della transizione ecologica è ovviamente in prima fila e il Ministero dello sviluppo economico funge da elemento di raccordo con il sistema industriale industriale e, in particolare, io richiamo sempre il sistema manifatturiero perché senza manifattura il Paese si siede economicamente.

su cui stiamo riuscendo a coinvolgere numerose realtà produttive del Paese e che permettono anche di superare quella che fino a oggi è stata una delle principali limitazioni a un intervento pubblico dello Stato per assecondare questa fase di transizione, cioè la disciplina degli aiuti di Stato. Fortunatamente - dico io - in questa fase, anche relativamente alla pandemia, la Commissione europea ha cambiato atteggiamento su questo. Non si è mai vista una grande fase di rivoluzione e riconversione industriale senza un accompagnamento, nei limiti dovuti, da parte dello Stato. Questo riguarda tutte le filiere industriali, alcune più esposte e altre meno. per quanto riguarda l'*automotive,* che lei ha richiamato nella sua interrogazione e su cui sto insistendo in questi giorni perché alcuni Paesi hanno già assunto decisioni e altri le stanno prendendo.

di euro e che ha come obiettivo il supporto alle piccole e medie imprese nella transizione ecologica digitale e innovativa; i contratti di sviluppo per 1,2 miliardi di euro a sostegno di programmi di investimento produttivi strategici e innovativi di grandi dimensioni;

oltre a tutto lo spiegamento di forze sul piano Transizione 4.0 e - mi piace ricordare - al nuovo bando macchinari innovativi, diretto ad agevolare le Regioni meno sviluppate e i programmi di investimento

superati dalla rivoluzione ambientale e digitale e che possono essere utilmente occupati nei nuovi settori che vengono avanti. Pertanto, si tratta di una sfida, che come ho già detto rispondendo a suoi colleghi, coinvolge davvero tutte le forze politiche, il Parlamento, il Governo e le forze sociali e su cui bisogna discutere e focalizzare di più l'attenzione. Purtroppo, però, la politica tendenzialmente si concentra sui piccoli interventi di breve termine.

In questo momento in Italia sono inesistenti gli incentivi per l'acquisto di autovetture ambientalmente compatibili (elettriche e non solo). Il mercato è totalmente fermo e io

e sussidiati da parte dello Stato. Tutti gli strumenti che ho ricordato (dai contratti di sviluppo a scendere) sono forme di intervento dello Stato in cui la risorsa pubblica può intervenire per una percentuale che è non totalitaria e neanche maggioritaria, ma comunque significativa in queste forme di investimento.

lei ha citato il maggiore ricorso al gas, ma non ho sentito una parola sul semplificare il *permitting* per le fonti rinnovabili, che sono la principale soluzione alla crisi energetica soprattutto delle aziende. Abbiamo presentato una mozione per dare più forza alle aziende e dare loro un credito di imposta sulle spese di autoproduzione energetica, perché dobbiamo puntare sul renderle il più indipendenti possibile. Non ho sentito dire una sola volta

una parola su uno dei principali strumenti per combattere la concorrenza sleale e incentivare gli altri Paesi a fare la transizione ecologica, ossia la *carbon border tax*, e il *carbon border adjustment mechanism*, che ne deve essere il meccanismo principale. Vorrei che il Governo si concentrasse maggiormente anche sulle speculazioni finanziarie, perché l'enorme tempesta di aumento di prezzi che abbiamo è certamente dovuta a situazioni oggettive (su questo non si discute), ma c'è anche una forte componente finanziaria di cui si parla